L’ordine del giorno reca: «Comunicazione, ai sensi dell’articolo 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di disegni di legge di conversione di decreti-legge». In data 18 agosto 2006 e` stato presentato il seguente disegno di legge: dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro per le politiche europee: «Conversione in legge del decreto-legge 16 agosto 2006, n. 251, recante disposizioni urgenti per assicurare l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione